Comunico che nella seduta di domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 18,30, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale renderà un'informativa sulla sicurezza nel Mediterraneo alla luce degli ultimi sviluppi. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori è convocata per la sua costituzione giovedì 27 maggio, alle ore 9, presso la sede di palazzo San Macuto.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

Senatori, desidero invitare quest'Assemblea a stringersi nel solenne ricordo del giudice Rosario Livatino in occasione della sua beatificazione come martire della giustizia e della fede. Nato a Canicattì nel 1952, Rosario Livatino era entrato in magistratura a soli ventisei iniziando immediatamente a occuparsi di criminalità mafiosa. Era un giudice coraggioso, capace, preparato; soprattutto, era un uomo fortemente legato ai valori della fede cattolica: valori vissuti anche attraverso il rigore della dedizione al lavoro, lo sforzo costante nella ricerca della verità in ogni fatto sottoposto al suo giudizio e la concreta attenzione alla persona, alla sua capacità di redimersi nonostante gli errori più gravi. Un giovane magistrato profondamente convinto che la giustizia avesse una funzione sociale imprescindibile e che fosse dovere del giudice applicare la legge con equilibrio e umanità. Una funzione che doveva essere misurata tanto sul piano della coerenza dell'azione giurisdizionale quanto su quello della trasparenza e dell'assoluta terzietà del giudice, condizione in cui egli credeva fermamente ricordando in più occasioni - con parole che acquistano oggi una nuova attualità come la credibilità esterna della magistratura nel suo insieme e in ciascuno dei suoi componenti rappresenti un valore essenziale in uno Stato democratico. Questo fu Rosario Livatino, un vero servitore dello Stato: autorevole, credibile e trasparente; un uomo innamorato della sua terra e determinato a difenderla, perseguendo instancabilmente verità e giustizia: quella Sicilia che nel pieno degli anni Ottanta viveva la sua notte più buia, lacerata dalle guerre di mafia, dalla corruzione e dalla spietata ferocia di un sistema criminale talmente compenetrato nel tessuto sociale da sembrare quasi impossibile estirpare. Un sistema che Rosario Livatino riuscì a contrastare con grande intelligenza. Fu tra i primi magistrati in Italia a fare ampio ricorso alla confisca dei beni come strumento per colpire al cuore la mafia, per depotenziarla, per dimostrarne la vulnerabilità, per far sì che non fossero più i cittadini a temere la mafia, ma che fosse la mafia ad avere paura dello Stato. E Rosario Livatino faceva paura a quella mafia spietata e vigliacca che la mattina del 21 settembre 1990 gli tolse la vita a colpi di proiettile in un feroce agguato, teso mentre si recava in tribunale senza scorta e a bordo della sua utilitaria. Una morte dolorosa per tutti, destinata a scuotere le coscienze non solo delle istituzioni e dei cittadini, ma di tutto il mondo cristiano. Indimenticabile è ancora nella nostra memoria quel «Convertitevi!», gridato nel ricordo anche di Rosario Livatino ai criminali mafiosi dall'allora pontefice San Giovanni Paolo II, proprio dalla Valle dei templi di Agrigento. La beatificazione - fortemente voluta da Papa Francesco - di Rosario Livatino come martire dei valori della Costituzione, sostenuti dalla forza di un'autentica fede cattolica, apre un nuovo importante capitolo nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Un capitolo in cui l'esempio e l'eredità morale di donne e uomini come Rosario Livatino può davvero guidarci verso un futuro sempre più libero dalle mafie, sempre più libero dalla corruzione, sempre più libero dalla violenza. *(Applausi)*.

Signor Presidente, è un onore per me poter commemorare in quest'Aula il beato Rosario Angelo Livatino. Le sue ultime parole furono «Picciotti, che cosa vi ho fatto?» e poi cadde sotto i colpi dei suoi sicari, e morendo li guardò in viso. Era il 21 settembre del 1990. Nelle sue parole troviamo l'eco delle parole del profeta Michea, che al capitolo 6 fa dire al Messia: «Popolo mio che male ti ho fatto? In che t'ho contristato?». Prima di consegnarsi alla morte, il Giusto chiese conto del male e così facendo restituì il rango di uomini a quelli che non erano diversi da bestie sanguinarie. Una delle cose che più mi ha colpito studiando la memoria di Rosario Livatino è che molti dei suoi sicari si sono convertiti in carcere, hanno abbandonato la mafia e hanno abbracciato la fede cristiana. Come ha già detto lei, signora Presidente, proprio tre anni dopo questo omicidio, il 9 maggio del 1993, in quelle stesse contrade echeggiarono le parole di san Giovanni Paolo II e non a caso il 9 maggio del 2021, quindi nella stessa data, il giudice Rosario Livatino è diventato beato. Rosario Livatino fu in prima linea contro la mafia, ma con sorprendente dote profetica seppe denunciare precocemente mali sociali che oggi, a trentacinque anni di distanza, si sono purtroppo mostrati in tutta la loro drammatica forza. Previde la deriva di una certa magistratura quando in un discorso tenuto il 7 aprile del 1984 disse: «L'indipendenza del giudice non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella sua conoscenza nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo dell'interferenza». Parole davvero profetiche. Previde e stigmatizzò anche i pericolosi esperimenti di ingegneria sociale con i quali oggi si mira a distruggere l'uomo e la famiglia, esperimenti oggi purtroppo all'ordine del giorno. Il 30 aprile del 1986 parlò chiaramente contro l'eutanasia, dicendo: «La posizione della morale cristiana sul punto è semplice e cristallina: essa si informa al principio dell'intangibilità, della sacralità dell'inviolabilità della vita umana». Parlò chiaramente anche contro la fecondazione assistita e l'utero in affitto, in quanto attività che potevano togliere al donatore la responsabilità di prendersi cura della discendenza, togliere ai figli la bellezza di conoscere il padre e la madre. Un uomo, un magistrato, un profeta e ora anche un beato: abbiamo bisogno di uomini come questi. Speriamo che dal Cielo interceda per noi.

e di riflettere sull'attualità del tema dell'impegno contro ogni forma di sopraffazione mafiosa, che inquina la vita economica, politica e sociale. Del resto, occasioni come questa assumono un significato tale si rifugge dalla retorica, diventano momenti per riflettere e occasioni per rinnovare la memoria dell'esempio di Livatino e del suo sacrificio, guardando al presente e al futuro, perché quei valori di legalità di libertà si proiettino nell'impegno cui ciascuno è chiamato ogni giorno. Il mese di maggio è purtroppo denso di anniversari, da quello della strage di Portella della Ginestra, del primo maggio di ai barbari omicidi di Pietro Scaglione e di Peppino Impastato, fino alla strage di Capaci. È impossibile non cogliere un legame proprio fra l'assassinio di Livatino e la purtroppo purtroppo lunga sequela di morti che insanguinarono i primi anni Novanta. Ho vivo il ricordo di quegli anni, del clima di paura, ma anche della capacità mostrata dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine, dalla scuola e dalla società civile, di saper reagire e di rispondere alla violenza mafiosa, non solo colpendo i responsabili, ma anche affermando la cultura della legalità, della legalità, intesa non solo come nome, per quanto doveroso, ma come rispetto delle norme e come corollario e condizione di libertà, libertà dalla paura e dal ricatto, libertà di vivere e di costruire, di pensare, di parlare e di fare impresa. A distanza ormai di una trentina d'anni da uno dei momenti più lunghi, nella lunga storia della Sicilia e del Paese intero, nel ricordare Livatino, al pari degli altri, tanti, troppi caduti nella lotta alla mafia, possiamo dire che quella stagione ha contribuito ad un profondo cambiamento culturale e al rifiuto da parte delle nuove generazioni del pesante retaggio mafioso. Diremmo oggi che Livatino era un ragazzo, o per meglio dire un giovane uomo, che semplicemente guardava al futuro, un futuro in cui, più che la mafia e persino l'antimafia, il rispetto delle leggi fosse la normalità. Da giurista attento, era capace di cogliere la delicatezza del ruolo di magistrato che ricopriva, attento a ribadire l'indipendenza della giurisdizione, ma anche i doveri connessi alla funzione. Valgono in tal senso, più di ogni altra cosa, le sue stesse parole. Infatti egli diceva che: «l'indipendenza del giudice (...) non è solo nella propria coscienza, nella (...) libertà morale, nella fedeltà

«nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni e in ogni momento della sua attività». Suona più che mai attuale il monito sull'esigenza di imparzialità, sostanziale e formale, di chi è chiamato a giudicare senza cedere alle sirene del protagonismo mediatico e anche in questo la lezione rappresentata dal pensiero e dalla stessa condotta di vita di Livatino offre lo spunto per riflettere, anche sul pericolo sempre attuale di strumentalizzazione dell'antimafia, di una sua trasformazione in professionismo. In questo, la profonda fede religiosa seppe accompagnarlo nell'affrontare il suo cammino, come qualcosa che completava e rafforzava la sua dedizione alla giustizia. Non è certo un caso che appena tre anni dopo, proprio nella sua stessa città...

anche noi del Gruppo Fratelli d'Italia vogliamo rendere omaggio in questa sede al giudice

Apolitico, autonomo e indipendente, lontano da condizionamenti di qualsiasi natura, ma anche pronto al dialogo e al rispetto di tutti gli attori del procedimento, non ultima certamente la persona da giudicare. Un uomo giusto, appunto un giudice, un magistrato col senso dello Stato, mai di parte. Non faceva interviste, Livatino; schivo nel carattere e del tutto privo di protagonismo, agiva con gli atti nei procedimenti, mai sui giornali. Un giudice come noi tutti vorremmo, e da cui noi tutti - ove mai accadesse - vorremmo essere giudicati. Anche se era considerato e definito «il giudice ragazzino», era in qualche misura un giudice all'antica, ma aveva nel contempo grande lungimiranza: fu tra i primi a prendere provvedimenti sul patrimonio dei mafiosi e a confiscarlo, sui colletti bianchi, sui reati contro l'ambiente e l'ecomafia; fu tra i primi a capire lo sviluppo del potere mafioso, la sua complessa articolazione anche politica, i conflitti interni, la guerra tra la stidda e la mafia. In tutto ciò, Livatino era certamente motivato anche dalla fede, da una fede incrollabile, e per questo anche ritenuto inavvicinabile. Nelle sue carte vi era sempre il riferimento semplice e diretto. Lui stesso scriveva: «Sotto la tutela di Dio»,

Credo sia importante sapere come Livatino sapesse coniugare perfettamente la sua fede, che lo motivava dal di dentro nelle sue azioni e lo rendeva incrollabile, con la necessità di applicare la legge dello Stato italiano. Siamo quindi orgogliosi, da cittadini italiani, da uomini delle istituzioni e da credenti, che sia anche riconosciuto come beato nel suo processo di santificazione, e che vi sia un giorno a lui dedicato: il 29 ottobre. In effetti, al di là della sua vicenda umana, ve n'è un'altra molto più significativa e pregnante che riguarda tutti noi sempre e comunque al di là delle generazioni, in cui nessuno di noi è giudice, anche se alcuni giudici pensano di esserlo comunque. Questa connessione in lui tra uomo di Stato e credente la si ritrova non solo nel suo comportamento da cittadino, e quindi da giudice, ma soprattutto negli accadimenti avvenuti dopo la sua morte e con la sua morte.

ma altri giudici agivano in quel contesto e non si fermarono. Come possiamo non ricordare la morte, nell'estate del 1992, prima del giudice Falcone e poi del giudice Borsellino in via D'Amelio? Come possiamo non ricordare la vedova Schifani che, nel sagrato della chiesa, da umile vedova del popolo disse: «Io vi perdono, però dovete mettervi in ginocchio»? Era quello un segnale chiaro di qualcosa di più forte dell'impegno civile.

Livatino, proclamato beato il 9 maggio. Non è una data casuale: è lo stesso giorno in cui il nostro Paese ricorda il rapimento di e l'omicidio di mafia di Peppino Impastato, due delle pagine più dure e dolorose della vita del nostro Paese. La Chiesa beatifica Livatino e, con un ennesimo gesto forte in Sicilia, conferma l'impegno dei cattolici contro le mafie e la distanza da quei mondi, che spesso cercano invece di usare la religione per crearsi consenso sociale. Rosario Livatino è stato il più giovane dei tanti magistrati martiri, vittime delle mafie; ucciso con terribile determinazione, in disprezzo della vita umana, in una vera e propria esecuzione. Perché? Perché - come recita la sentenza di condanna dei mandanti ed esecutori del delitto - «perseguiva le cosche (...)

era un uomo che faceva il proprio dovere. Aveva perseguito e fatto condannare gli uomini della stidda; aveva avuto il coraggio di applicare in modo innovativo ed efficace - come ha ricordato il Presidente - le misure di prevenzione. Fu il primo a trovare il modo di confiscare i beni dei mafiosi. Sapeva dei rischi che correva nella Sicilia delle guerre di mafia, ma proprio per questo, per non mettere in pericolo altre vite (ricordiamolo), rifiutò la scorta e si trovò da solo di fronte ai suoi esecutori. La sua bravura, la sua determinazione non gli hanno mai fatto, però, perdere di vista l'umanità; non ha mai concepito l'azione penale come vendetta ed è arrivato a perdonare i suoi assassini. Rosario Livatino teneva al suo lavoro, si batteva per il rigore e la credibilità della magistratura. In un ambiente difficile, ha scelto di stare là dove stava il nemico più pericoloso, la mafia, e non si è mai arreso e non ha mai arretrato. Facendo il suo dovere, non ha mai smesso di testimoniare la propria fede. Oggi ricordiamo un uomo che è un esempio; deve esserlo, come cristiano, come uomo e come magistrato. Ma voglio anche ricordare in questa occasione un uomo, Piero Nava, che ha avuto il coraggio di denunciare, identificare e testimoniare al processo, facendo sì che gli esecutori di quell'orrendo delitto fossero puniti. Piero Nava ha fatto una scelta di civiltà e di senso civico che ha cambiato la sua vita; ma ci ha detto - nelle interviste in questi mesi, dopo anni - che è orgoglioso di quella scelta. Io credo che oggi facciamo bene a ricordare in quest'Aula per dire che le istituzioni non dimenticano chi ha saputo rappresentarle così bene, chi ha saputo rappresentare lo Stato e il Paese, arrivando fino all'estremo sacrificio. Grazie quel 21 settembre del 1990 la notizia dell'uccisione di Rosario Livatino mi giunse mentre mi trovavo a Roma alla Commissione parlamentare antimafia come consulente. Tornai immediatamente a Palermo, raggiunsi in procura Giovanni Falcone, che già si era insediato come procuratore aggiunto, e insieme, addolorati e sgomenti, cercammo di comprendere le ragioni di quel vile attentato. Sapevamo che come pubblico ministero si era occupato della prima rilevante indagine sulla mafia agrigentina che aveva portato alla condanna di molti mafiosi. Riferii a Falcone che lo avevo incontrato a maggio, pochi mesi prima, in occasione di una missione della Commissione antimafia al tribunale di Agrigento decisa dopo uno sconvolgente susseguirsi di omicidi che, per la loro efferatezza, avevano colpito l'opinione pubblica. Da circa un anno era passato come giudice allo stesso tribunale ed era stato destinato alle cause civili, ma per le note carenze di magistrati si occupava a tempo pieno di misure di prevenzione e confische di beni. Il giorno dopo andai con Falcone ai suoi funerali a Canicattì. Ho ricordi vividi di quel momento: la bara portata a spalla dai suoi colleghi, deposta in chiesa, avvolta dalla toga e dal Tricolore, coperta di fiori; accanto, in piedi, sei magistrati in toga; dietro, due corazzieri inviati dal Presidente della Repubblica. Una forte ondata di emozione pervase il Paese, che solo in quel momento scoprì la sua storia di uomo buono, la sua vita di giudice rigoroso e schivo, il suo volto pulito. Diventò per tutti e sarà per sempre il giudice ragazzino. È importante ricordare quanto fosse pesante in quel momento l'atmosfera in Sicilia, perché emerge con ancora più forza il suo coraggio, il suo diventare suo malgrado un martire. Grazie all'immediata collaborazione di un testimone oculare, Pietro Nava, che sarà costretto, per la sua sicurezza, ad abbandonare il lavoro di agente di commercio e ad emigrare all'estero, le indagini e tre processi susseguitisi negli anni hanno fatto piena luce sulle cause, sui mandanti, sugli esecutori di quell'eccidio. Quella tiepida mattina del 21 settembre 1990, riposti nella borsa i fascicoli studiati fino a tarda notte dell'udienza delle misure di prevenzione, che voleva definire dopo aver addirittura rinviato le ferie, percorreva come ogni mattina a bordo della sua autovettura la superstrada che da Canicattì lo portava al tribunale di Agrigento, quando un commando di quattro uomini gli sbarrò la strada e aprì il fuoco. Ferito a una spalla, una pistola si inceppò, lui fuggì a piedi, ma venne braccato come una preda, inciampò, si fratturò una caviglia e quando venne raggiunto in fondo alla scarpata, all'inseguitore pose la domanda di chi ha sempre agito secondo coscienza: picciotti, cosa vi ho fatto? La risposta fu un colpo di grazia alla testa. Un'eliminazione, la sua, compiuta da *killer* di Palma di Montechiaro e di Canicattì quale espressione della lotta congiunta a cosa nostra da parte di gruppi criminali emergenti, i componenti della cosiddetta stidda che volevano dimostrare, con l'uccisione di un giudice, la loro potenza criminale. Su una pagina della sua agenda e in altri suoi scritti si rinvenne una piccola croce e sotto la sigla STD; le tre lettere furono un vero rompicapo; la spiegazione si trovò nella sua tesi, nella sua fede: *sub tutela dei,* invocava l'assistenza divina nella sua opera di giudice. Egli aveva una fedeltà alla legge e alla propria coscienza, un impegno alla preparazione professionale, un'estrema cura nelle decisioni, una rigorosa condotta di vita, serietà, equilibrio, responsabilità, umanità, quella di cui ancora oggi la magistratura dovrebbe dare testimonianza quotidiana per togliersi quell'ombra di sistema correntizio e di potere politico, mediatico e giudiziario che, a causa del comportamento di alcuni suoi componenti, infanga la credibilità di un'intera categoria.

annunciando che la Commissione parlamentare antimafia ha poco fa approvato all'unanimità una relazione, che sarà inviata a entrambe le Camere, illustrativa del contesto criminale in cui è maturata l'uccisione di Rosario Livatino, nonché del suo ruolo e dei suoi provvedimenti, per dare un quadro completo sull'esemplare opera di questo magistrato.

2021 è beato. La Chiesa cattolica lo venera come martire di giustizia. Livatino è un esempio di piena coerenza tra fede, vita e professione di magistrato. Ne riscontriamo il percorso coerente sin da quando, negli anni del liceo, si impegnò nell'Azione cattolica, nella preghiera e nella diuturna visita al Santissimo Sacramento - tanto che i mafiosi lo definivano spregiativamente "santocchio" e in un primo tempo, per tale ragione, pianificarono l'agguato davanti alla chiesa - nonché nella quotidianità di vita e di attività professionale. Basti pensare che su tutti gli appunti, i documenti, i quaderni era riportato l'acronimo STD, che gli investigatori, dopo la morte, impiegarono tempo per decodificare, ma che voleva dire *sub tutela Dei.* Il suo impegno professionale lo ha portato anche a riflettere e approfondire le caratteristiche del magistrato e il dovere di non piegare la legge all'interesse di parte. Ancora, sul rapporto fra magistrato e politica, nel 1984 diceva: «Sarebbe sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l'ufficio del giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi dietro tutti i vascelli alle spalle, con le dimissioni definitive dall'ordine giudiziario». Nel 1986 rifletteva su regole valide per chiunque eserciti la giurisdizione: «Il compito del magistrato è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere numerose cose o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata». Nell'agenda di Livatino il 18 luglio 1978 è annotato: «Oggi ho prestato giuramento; da oggi sono in Magistratura». «Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige». Scusate l'emozione, ma ho conosciuto proprio in quell'anno Rosario Livatino, che frequentava il corso sul diritto della persona e del diritto di famiglia che tenevo come componente del Consiglio agli uditori giudiziari. *(Applausi)*. È stata enorme, poi, la tragedia ai miei occhi, quando alcuni anni dopo la sua morte, andando nella sua casa, sulla sua scrivania ho trovato un *bloc-notes* di appunti su quelle lezioni, con il mio nome impresso sulla prima pagina. Livatino entrò in magistratura nel 1978 e dal 1978 al 1979 fu pubblico ministero ad Agrigento. In quel periodo si è occupato di processi di mafia, ma anche di criminalità comune. Dal 1989 passò invece alla giudicante come giudice *a latere* per occuparsi - come è stato già ricordato - di sequestri e confische di beni. Morì come aveva vissuto, rispettando gli imputati, anche quelli che si erano macchiati dei più gravi delitti perché erano innanzitutto persone: era questo il suo credo. *(Applausi).* A volte andava all'obitorio a pregare davanti al cadavere dei mafiosi uccisi. Una volta, in un caldissimo ferragosto, portò personalmente in carcere il provvedimento di scarcerazione di un recluso. A chi si stupiva disse: «All'interno del carcere c'è una persona che non deve restare neanche un minuto in più. La libertà dell'individuo deve prevalere su ogni cosa». non so ancora come pregarti e chiederti aiuto, ma ti chiedo di illuminare noi tutti nell'individuare le riforme giuste per una giustizia come la intendevi tu. *Vale* Rosario.

come faceva tutti i giorni, senza scorta; parole forti di un'innocenza che ha ferito - come sappiamo - anche i suoi carnefici. un giudice che affrontava i mali in tutti i suoi aspetti, per salvare le vittime e i colpevoli; un uomo che ha perseguito una verità, una sola, quella della giustizia e lo ha fatto a costo della sua stessa vita, come un pazzo, come un sognatore, perché senza pazzi e sognatori non ci sarebbe futuro. Rosario Livatino camminava per le strade di quella Sicilia malata di silenzi, di sottomissione, di teste chine da parte di chi doveva lottare per la giustizia, ma cedeva alla paura. Rosario invece non si nascondeva, camminava senza scorta, consapevole di essere nelle mani di Dio e dicendo una cosa importante, una grande verità: «Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». La sua credibilità stava in un'immensa fede in un'immensa fede tanto nel Signore quanto nella libertà; libertà, giusto motore delle nostre azioni, che può essere però rischiosa. Eppure, nessuna esistenza può prescindere dalla libertà e noi tutti dobbiamo fare tesoro di vite così concrete da far venire i brividi anche anche alle mafie peggiori, a tutte le mafie del mondo, anche se sul selciato della libertà sono caduti preti, magistrati e avvocati; vite che guardavano in faccia i colpevoli perché alla ricerca dell'uomo, alla ricerca dell'anima, gente che andava oltre il reato. Così faceva Rosario: non abbassava lo sguardo davanti ai colpevoli durante i suoi giudizi e piangeva davanti alle loro uccisioni. E allora il sangue versato da lui e dagli altri martiri va a dissetare una terra meravigliosa, ma malata, perché le mafie - mie care senatrici, miei cari senatori - sono lì, sono qui e noi abbiamo il dovere di trasformare il sangue versato in azioni concrete, in leggi dello Stato, in modelli da seguire per i nostri figli e nipoti. Rosario quel 21 settembre 1990 perde la vita e oggi è il primo magistrato nella storia a diventare beato. *Sub tutela dei*: c'era scritto nell'agenda trovata vicino al suo corpo senza vita. È infatti nelle mani del Signore che è stato consegnato quel 21 settembre del 1990 ed è nelle sue mani che resterà per sempre.

delle elezioni e delle immunità parlamentari secondo la previsione dell'articolo 68 della Costituzione.

querelanti Rocco Giacomazzi e Lucio Massimo Marino di Telesud 3 srl. L'ho però cancellato dalla discussione perché il tribunale di Trapani, con sentenza del 30 aprile 2021, n. 517, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del senatore Santangelo per estinzione del reato a seguito di remissione della querela.

n. 1, per declaratoria di insindacabilità avanzato dalla senatrice Anna Maria Bernini, pendente presso l'organismo di mediazione forense di Roma; n. 2, per declaratoria di insindacabilità avanzato dal senatore Franco Mirabelli, pendente presso l'organismo di mediazione forense di Roma.

e un altro nei confronti dello stesso senatore Armando Siri, relativamente a un procedimento penale ancora pendente presso il tribunale di Milano. A questo proposito voglio far presente che, con provvedimento del tribunale del riesame del 19 maggio 2020, è stato annullato il decreto di sequestro emesso nei confronti del signor Luca Perini, collaboratore del senatore Siri, e tale annullamento è stato confermato dalla Corte di cassazione nell'udienza dell'8 ottobre 2020. La procura di Milano ha scritto in data 18 maggio 2021, ritenendo ancora attuali entrambe le richieste di autorizzazione relative al senatore Siri in relazione alla mutata qualificazione giuridica delle condotte, ferma restando l'identità dei fatti materiali. Su questo ha chiesto la parola il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

documento n. 3, nei confronti dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi (procedimento penale pendente presso il tribunale di Bologna); nei confronti del senatore Luigi Cesaro (procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli); il documento n. 8, nei confronti del senatore Roberto Marti (procedimento pendente presso il tribunale di Lecce).

la Giunta per il Regolamento, riunitasi l'11 maggio 2021, ha espresso il seguente parere: «Tenuto conto della disciplina prevista per i Gruppi parlamentari dall'articolo 14, comma 4, terzo periodo, del Regolamento, è consentita la costituzione di componenti politiche all'interno del Gruppo Misto purché rappresentino partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali. I senatori che intendono costituire una componente politica all'interno del Gruppo Misto devono essere autorizzati a rappresentare il partito o movimento politico detentore del contrassegno presentato alle elezioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di tale formazione politica. Per le dichiarazioni di voto finali del Gruppo Misto, la Conferenza dei Capigruppo stabilisce i tempi aggiuntivi previsti dall'articolo 109, comma 2-*bis*, del Regolamento e i tempi assegnati ai senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni espresse dal rappresentante del Gruppo Misto.

quella dove dice che anche per le componenti occorre riferirsi a un Gruppo. Ovviamente noi non siamo d'accordo e troviamo liberticida questa interpretazione; ma è chiara

Senatore Crucioli, forse la mascherina non ha fatto sentire bene le espressioni che ho appena letto, che sono il frutto di una decisione della Giunta per il Regolamento. Per quello che riguarda la regolamentazione del dissenso, lei sa che c'è un comma primo dell'articolo 109 - che sarebbe poi un secondo, perché il primo è stato abrogato, se non ricordo male - che regola il dissenso di tutti i Gruppi parlamentari.

per il dissenso si farà egualmente. Si assegnerà un tempo anche per il dissenso rispetto a quella che è la dichiarazione di voto del Gruppo Misto. È chiaro? Forse detto in questo

esaminare il disegno di legge n. 2201, di conversione del decreto-legge n. 42

Il decreto-legge del Governo Draghi pone correzione e, anzi, impedisce che si formi una falla nel sistema della sicurezza alimentare, così come previsto e voluto, forse per svista, per errore o per un diverso disegno o una diversa intenzione politica, dal precedente Governo Conte II. Mi riferisco, in particolare, del decreto legislativo n. 27 del 2021. Con questo decreto legislativo, dal giorno 26 marzo sarebbero

contravvenzionali e sanzioni amministrative che costituiscono il tessuto sul quale è formato parte del sistema dei controlli che attengono alla sicurezza alimentare. Come sappiamo, c'è una prima fascia più importante di delitti che attengono alle contraffazioni e alle sofisticazioni alimentari

di non doversi procedere perché il fatto non è più reato e non ha più alcuna conseguenza, con l'ulteriore caratteristica che in quel caso il giudice, davanti a un'eventuale contravvenzione, non avrebbe neppure segnalato alle competenti autorità amministrative

Governo voleva introdurre una nuova visione ispirata dall'Europa. Tutto discende dal fatto che la normativa europea e la legge delega del 2019 attribuiscono agli Stati un compito di rivisitazione

consentire il mantenimento delle sanzioni penali, quindi dei controlli a tutela della sicurezza alimentare. In sede di conversione alla Camera sono stati introdotti anche due articoli molto importanti: il primo sostanzialmente costituisce una garanzia difensiva, cioè la possibilità di estendere l'articolo 223 del codice di procedura penale (disposizioni attuative), cioè di essere informati nel momento in cui si svolgono indagini, anzi nel momento in cui si stanno svolgendo analisi sui campioni dei prodotti oggetto di inchiesta per eventuale contraffazione

sede di conversione alla Camera, consente di rendere non applicabili le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 91 del 2014 qualora vi sia un ravvedimento operoso. Pongo

a questa norma perché di fatto consente, a chi si mette in regola entro giorni - e non più novanta - dalla cosiddetta diffida, di evitare la sanzione amministrativa. Si tratta di una norma di buonsenso, non punitiva, che tiene conto anche delle diverse esigenze che possono esserci nel mondo della produzione nel settore agricolo.

che impedisce che il nostro sistema si trovi aperto a insidie improvvise per mancanza di una normativa che sarebbe stata cancellata di fatto

Signor Presidente, l'industria alimentare italiana di cibi sia di produzione che di trasformazione è tra le migliori sul mercato internazionale. L'attenzione verso questo settore è essenziale, in considerazione dell'importanza che tale industria manifatturiera riveste nel nostro sistema economico-sociale. Infatti, l'Italia è il Paese dove si sono creati i prodotti diventati oggi il nostro patrimonio conosciuto e rispettato da tutto il mondo: il *made in Italy* agroalimentare. Non possiamo far venir meno la *leadership* raggiunta a livello internazionale e dobbiamo mantenere altissimo lo *standard* di sicurezza dei nostri prodotti alimentari. Non dimentichiamo che la sicurezza alimentare ha caratteristiche di bene pubblico; occorre garantire livelli di sicurezza a beneficio del consumatore e della salute pubblica. In tale direzione va la corretta tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle materie prime da cui derivano. La corretta tracciabilità è il pilastro delle politiche per rendere trasparente la scelta dei cibi, in considerazione anche del fatto che vediamo crescere nei consumatori sempre più alte aspettative. Qui si tratta di un controllo che riguarda prodotti italiani o di altra provenienza destinati a essere commercializzati sul territorio nazionale o destinati ad altri Stati dell'Unione o anche esportati. Lo scopo del controllo è fornire ai consumatori informazioni accurate sui prodotti e garantire la circolazione di alimenti sicuri, grazie alla possibilità di ricostruire l'intero percorso degli alimenti per poter ritirare tempestivamente - se è il caso - quelli a rischio. Questo sistema complesso di controlli si svolge su tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione, magazzinaggio, trasporto e commercio e della somministrazione. Il decreto in sede di conversione è finalizzato a correggere l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che dà seguito al regolamento europeo che abrogava inspiegabilmente diversi illeciti. Perciò il decreto in esame è finalizzato a evitare che rilevanti settori restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, esponendo così a gravi rischi per la salute dei consumatori Per Forza Italia la sicurezza alimentare è stata sempre motivo di grande attenzione: lo dimostra la battaglia in Europa del Governo Berlusconi dal 2002 per ottenere la sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare a Parma

Purtroppo lo stesso impegno per avere in Italia una sede dell'Agenzia del farmaco, l'EMA, non è stato profuso da Governi recenti, non votati dagli italiani, perché in Europa si deve lavorare prima

perdendo così la possibilità di crescita del PIL del 2 per cento. Le nostre leggi nazionali in tema di sicurezza alimentare sono le più rigorose in Europa e forse nel mondo e questa giusta sicurezza per la salute dei nostri cittadini ovviamente ricade sui nostri prodotti che hanno costi di produzione superiori ai Paesi concorrenti. Il mio appello al Governo è che si faccia promotore in Europa di un adeguamento degli altri Paesi alle nostre leggi sul tema della sicurezza alimentare. Invito anche tutti i parlamentari europei a sostenere la battaglia di Forza Italia contro l'abominio del nutri-score, l'ultima trovata del vino annacquato, l'etichettatura anticancro dei salumi, eccetera. Confido nella difesa di questo Governo e invito i parlamentari europei degli altri Gruppi politici ad essere più presenti nelle Commissioni di merito per difendere gli interessi del Paese senza altre bandiere che quella italiana, come fanno gli altri, e a dialogare di più con i parlamentari nazionali, affinché non ci arrivino sul tavolo regolamenti ormai immodificabili. *(Applausi)*.

e quella del Gruppo al quale appartengo in relazione al presente decreto-legge che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Mi sono personalmente fatto carico della questione oggetto del decreto-legge insieme ai colleghi della Commissione agricoltura, interagendo proprio con il Ministero, al fine di porre riparo alla situazione grave che si sarebbe determinata in assenza di una tutela penale e amministrativa nella materia alimentare. Il provvedimento, infatti, circoscrive l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. che per l'appunto avrebbe comportato l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi, di cui alla legge n. 283 del 1962, proprio in materia di sicurezza alimentare. La legge n. 283 del 1962 reca la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo tra l'altro numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica. Essa costituisce il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare rispetto ai più gravi delitti previsti dal codice penale, *ex* articolo 439 e seguenti, applicabili quando gli eventi si sono già verificati. La normativa vieta la vendita, la somministrazione e l'impiego di alimenti e bevande private, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali, con l'aggiunta di additivi chimici, di qualsiasi natura, non autorizzati con decreto del Ministero della salute o, nel caso siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. Quindi, si può ben capire l'importanza della reintroduzione di questa normativa. Dalle predette violazioni discende la pena dell'arresto e dell'ammenda, variamente determinata. Dunque il decreto-legge in esame evita che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restino privi di tutela sanzionatoria, penale e amministrativa, in risposta alla inaspettata depenalizzazione, introdotta con il decreto legislativo n. 27 della quale peraltro non vi era traccia nello schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento per il prescritto parere e che avrebbe potuto presentare anche un possibile vizio di eccesso di delega, come affermato anche dalla Corte di cassazione, ufficio del massimario, nella relazione del 17 marzo 2021. La legge di delega, infatti, prevedeva soltanto la possibilità di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625, con l'abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili, oltre a conferire al Governo soltanto il potere di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE

ed esponente del MoVimento 5 Stelle, che ha sempre avuto a cuore le tematiche ambientali e alimentari, e primariamente come cittadino, ritengo che l'elevata tutela prevista per il consumo e il commercio di prodotti di qualità sia essenziale, sia per dare effettiva applicazione al diritto alla salute, sia per proteggere la qualità dei nostri prodotti. Il presente decreto-legge contribuisce a ripristinare e a implementare le finalità

leggere le premesse al disegno di legge in esame, che ci apprestiamo a votare oggi, in seconda lettura. Leggo testualmente alcuni passaggi, a mio avviso significativi: «l'intervento normativo è urgente, ha lo scopo di evitare che si produca l'abrogazione di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo, previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283» Salto alcuni passaggi di carattere tecnico e continuo sempre a leggere testualmente: «Senza questo intervento, che evita l'abrogazione delle fattispecie di illecito penale e amministrativo, si produrrebbe l'effetto di lasciare del tutto privi di tutela alcuni settori importanti per la salute dei consumatori, effetto certamente non voluto, quantomeno perché non previsto dalla legge di delega, in forza alla quale è stato adottato il decreto legislativo n. 27 del 2021 e non accompagnato, nel medesimo decreto legislativo, da interventi di natura sanzionatoria idonei ad incidere sui medesimi ambiti». In sostanza, cari colleghi, si dice in maniera anche molto esplicita, che bisogna mettere una toppa all'errore fatto dal precedente decreto, con cui si eliminava tutta una serie di norme sanzionatorie a tutela del consumatore e non solo. Attenzione, quindi: questo non lo dice il senatore La Pietra di Fratelli d'Italia perché è all'opposizione e quindi in qualche modo dobbiamo trovare qualcosa da contestare, ma lo scrive il Governo nella prefazione del disegno di legge. Già di per sé, quindi, credo si dovrebbe stigmatizzare questo fatto, ma soprattutto si dovrebbe capire da dove e da chi nasce questo errore macroscopico dell'aver cancellato quelle norme sanzionatorie. È stato solo un errore, una svista di per sé già grave, oppure c'è stata la famosa manina che in qualche modo - e non si capisce come - all'insaputa di tutti è riuscita a scrivere questa cosa? Non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai; fatto sta che molto spesso abbiamo riscontrato che questa manina ogni tanto appare e stravolge quanto scritto nei decreti. Non è la prima volta e forse non sarà l'ultima, purtroppo.

tornando al merito, è chiaro che questa svista - chiamiamola così per essere benevoli -, fatta salva comunque la tutela della salute dei consumatori, avrebbe aperto una serie di situazioni che - attenzione - non avrebbero avvantaggiato i nostri agricoltori e produttori,

è certo l'obiettivo principale della produzione. In sostanza, sarebbe stato un danno irreparabile per le nostre produzioni agroalimentari di qualità, e avrebbe aperto il mercato a prodotti che non mi perito a considerare e definire prodotti spazzatura. Colleghi, forse non ci sarebbe da parlare molto su questo provvedimento, poiché si tratta fondamentalmente di tre articoli complessivi, di cui solo il primo è sostanziale; quindi poco c'è da dire. Ma lascio queste considerazioni al al collega Balboni, che meglio di me saprà entrare negli aspetti tecnico-giuridici. Quello che mi meraviglia è che abbiamo parlato comunque poco delle conseguenze e dell'impatto di questa norma sia sulla sicurezza alimentare, sia sulle nostre produzioni di eccellenza. Ripeto, non per generare incomprensioni, che la salute dei consumatori è per noi prioritaria, ma è anche di fondamentale importanza tutelare i nostri prodotti agroalimentari con leggi severe, e siamo convinti che anche le pene devono essere severe. Quindi, tutela dei produttori e dei consumatori: lo dico perché, quando ci troviamo di fronte ad una frode alimentare, non c'è solo un danno diretto e specifico del prodotto in questione, ma molto spesso c'è un danno generale a un'intera filiera o a un intero comparto. Credo che tutti noi ricordiamo lo scandalo del vino al metanolo o i recenti scandali sulla pasta, e potremmo citarne altri. è che queste frodi non danneggiano solo chi le compie, ma danneggiano l'immagine di tutto un settore che non può permettersi sbagli di questo tipo. Chi sbaglia deve essere punito, e per noi si dovevano addirittura inasprire ancora di più le sanzioni verso coloro che danneggiano con il loro comportamento l'immagine della qualità italiana: lo consideriamo né più e né meno alla stregua di un vero e proprio tradimento. Ma se da una parte diciamo che chi sbaglia deve pagare e che le pene siano anche più severe, dall'altra diciamo anche che il Governo deve mettere in campo politiche che aiutino i nostri agricoltori, i nostri allevatori e i nostri pescatori; politiche che devono avere due obiettivi fondamentali, uno complementare all'altro. In primo luogo, occorrono maggiori tutele per i marchi italiani contro le contraffazioni che tolgono alle nostre aziende un potenziale mercato che vale più del doppio delle nostre esportazioni. a fronte di circa 50 miliardi di esportazione dell'agroalimentare, ci sono oltre 100 miliardi di falsi prodotti italiani (il fenomeno dell'*italian sounding*). E qui il nostro Governo dovrebbe essere forte nel chiedere maggiori tutele, soprattutto sul fronte interno europeo; così come dovrebbe essere più forte e determinato nel chiedere l'abolizione di sistemi di certificazione della qualità che penalizzano i nostri prodotti di eccellenza rispetto a quelli spesso fatti in laboratorio: mi riferisco al nutri-score, il sistema di etichettatura a semaforo; dovremo effettivamente discutere della sua valenza sul piano della buona alimentazione. Occorre maggiore attenzione alle dinamiche relative all'importazione di prodotti dall'estero che sono palesemente di scarsa qualità, ma che, per i meccanismi di rimbalzi internazionali, entrano nel mercato europeo e danneggiano i nostri produttori. Se vogliamo fare un esempio recente, basti pensare al miele cinese, fatto con sciroppi zuccherati e che entra nel mercato con prezzi ridotti dell'80 per cento rispetto al prezzo medio di un normale miele naturale.

quindi, tutela dei nostri prodotti; ma poi, come secondo elemento, occorrono politiche economiche e finanziarie per aiutare l'agricoltura. Occorre tutelare il reddito degli agricoltori. Spesso, nelle filiere agroalimentari, gli attori a monte e a valle della filiera, cioè i produttori e i consumatori, sono i più penalizzati: si parte da prezzi sempre più bassi, che rischiano di strozzare i produttori, per poi arrivare al consumatore, con prezzi spesso dieci volte maggiori del prezzo pagato alla fonte. alla fonte. La grande distribuzione deve farsi carico dell'onere di valorizzare maggiormente il lavoro degli agricoltori. Occorrono, poi, risorse per investire in tecnologia e regole per facilitare le procedure finanziarie, dirette ad agevolare il credito agli imprenditori agricoli. In Italia abbiamo un parco di macchine agricole ormai vecchio e poco produttivo, senza parlare della flotta peschereccia, ormai obsoleta per la stragrande maggioranza delle imbarcazioni. Maggiori investimenti significano anche migliore qualità e maggiore sicurezza alimentare. Ci sarebbe ancora molto di cui parlare, signor Presidente, ma voglio concludere citando un altro elemento importante, che riguarda i controlli. Abbiamo bisogno di più controlli sui prodotti che arrivano nel nostro Paese e, soprattutto, di ridurre gli accessi portuali per un controllo più capillare. Contemporaneamente, però, abbiamo bisogno di una semplificazione di tante procedure, che spesso soffocano le nostre aziende agricole, che hanno un solo e unico interesse: produrre qualità e sicurezza alimentare. qualità e sicurezza alimentare. Infine, occorre prendere spunto da quanto accaduto con questo provvedimento per fare una riflessione profonda su cosa significhi la sicurezza alimentare e soprattutto sulla normativa che ne definisce confini,

forse ad un testo unico, più adeguato ai nostri tempi e che contemporaneamente, da una parte, consenta una maggiore tutela della salute dei consumatori e, dall'altra, cerchi di agevolare, snellire e meglio controllare questo importante settore dell'economia nazionale che è l'agroalimentare. *(Applausi)*.

Tutta la rocambolesca vicenda, che a grandi linee poi accennerò, è lo specchio della confusione che negli ultimi mesi sta vivendo la politica italiana. Infatti, questa confusa vicenda ci deve interrogare sulle modalità di svolgimento dei lavori legislativi, nella fattispecie in una materia così delicata quale è quella della sicurezza alimentare. Il decreto-legge che ci apprestiamo il decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021

su una materia importantissima relativa al controllo della sicurezza degli alimenti. Il decreto legislativo n. 27 del 2021 (quindi il primo) doveva disporre l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione europea n.

che fissava i principi e i criteri direttivi specifici per l'adeguamento con uno o più decreti legislativi della normativa nazionale in tema di controllo ufficiale in materia di alimenti e bevande. quindi uniformarla al succitato regolamento europeo. Tuttavia, con probabile e quasi certo vizio procedurale di eccesso di delega, rilevabile previo promovimento di incidente di costituzionalità in via incidentale in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in ragione del mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi specifici impartiti dal Parlamento, l'articolo 18, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 27 del 2021 andava a abrogare la legge n. 283 del 1962 e tutte le successive modifiche,

Nel frattempo si insediava il nuovo Governo che, sollecitato sull'argomento anche e soprattutto dalla dottrina (possiamo vedere la relazione del massimario della Cassazione n. 13 del 17 marzo 2021)

non ha abrogato le disposizioni abrogative della legge alimenti contenuta nel decreto legislativo n. 27 n. 27 del 2021, ma ha preferito mantenere l'abrogazione e ha recuperato gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 22, nonché quelli correlati alla legge di modifica n. 441 del 1963 e al relativo regolamento di esecuzione, salvando così, almeno in calcio d'angolo, gli illeciti con relative sanzioni. Restano però alcuni interrogativi, come ha detto qualche collega che mi ha preceduto. Per esempio, le disposizione contenute nel decreto legislativo n. 27 da dove arrivano? Non erano contenute nella bozza di decreto-legge varato dal Governo il 20 ottobre 2020, diramato dall'Esecutivo alle Commissioni parlamentari per i pareri prescritti. È quindi lecito chiedersi chi realmente ha tentato di abrogare le disposizioni preventive a tutela della salute dei cittadini in un campo così importante come la sicurezza degli alimenti. Soprattutto però emerge quanto sia importante un sano ed adeguato controllo politico su quanto viene proposto sotto lo schema di inesistenti esigenze tecniche per far passare contenuti a volte anche pericolosi per i cittadini. In merito avevo presentato anche una interrogazione al ministro Patuanelli, subentrato

ad inserire nel parere almeno l'orientamento del regolamento dell'Unione europea, che era quello di perseguire una intenzionale di depenalizzazione della contravvenzione alimentare, con contestuale sua trasformazione in illecito amministrativo. In questo parere, che ha avuto poi l'unanimità della Commissione, è stato inserito anche che, oltre a recuperare l'abrogazione di alcune norme contenute nella legge del 1962, potevamo fare qualcosa di più, ma ci riserviamo di farlo al prossimo provvedimento utile. Concludo affiancandomi alla richiesta di Federconsumatori del 22 marzo: per evitare per evitare che in futuro accadano simili episodi, si chiede al Governo - e investo di questa richiesta istituzionale il Governo - di istituire al più presto un tavolo sulla sicurezza alimentare che veda come protagoniste le associazioni dei consumatori.

Italy.* Già il provvedimento merita il voto favorevole perché va a sopperire a una pericolosa lacuna che si era creata,

e nell'esclusivo interesse del settore. Restano comunque aperti quegli interrogativi che prima o poi andremo a verificare. *(Applausi)*.

credo vada sottolineato prima di tutto un aspetto, cioè che la salute pubblica, con riferimento alla sicurezza alimentare,

depenalizzando di fatto una serie di illeciti, ha posto comunque rimedio con sollecita immediatezza il Governo attualmente in carica. *(Applausi)*. Vorrei dirlo perché, al di là di quelle che possono essere le dietrologie del caso, visto e considerato che comunque siamo insieme, almeno dovremmo capire è stato una cosa buona fatta dal presidente Draghi e dal ministro della giustizia Cartabia, tra l'altro in un periodo come marzo, in cui c'erano molte gatte da pelare,

oppure in cattivo stato di conservazione, oppure con microbi di vario genere come additivi chimici, oppure per la vendita di alimenti insudiciati con parassiti, alterati, tossici. Era stata anche tolta la possibilità di chiudere gli stabilimenti e non era più considerata illecita, ad esempio, l'omissione di determinate indicazioni importanti

da dove nasce il pasticcio può interessare o meno, però il punto fondamentale è che è stato presentato un decreto-legge, quindi con la massima urgenza, per evitare che questa

Signor Presidente, Governo, colleghi, dedico questi minuti non solo all'ennesimo regolamento da applicare, ma ai produttori italiani che devono esercitarlo, a loro che devono sempre rispettare ciò che viene chiesto dalla politica italiana e soprattutto europea. Nel comunicare questa opportuna variazione legislativa, faccio notare che per gli operatori del settore alimentare e mangimistico, all'articolo 1-*bis* sono reintrodotte le garanzie in materia di analisi dei campioni e si tornano ad applicare le norme che danno la possibilità agli operatori di partecipare con un esperto all'esecuzione della prova delle analisi. All'articolo 1-*ter* finalmente si introduce l'istituto della diffida in materia di sicurezza alimentare, che permette agli operatori del settore alimentare di sanare violazioni dovute a semplici errori o omissioni formali. All'articolo 3 si richiede la pubblicazione di caratteristiche, modalità e risultati in un piano di controllo nazionale pluriennale, atti a valutare l'efficacia e l'efficienza anche della pubblica amministrazione. Agli articoli 7 e 8 si danno indicazioni per l'applicazione dell'istituto della controperizia e controversia documentale e analitica. Nel nostro Paese queste non sono tutte una novità, ma vanno a sostituire la ripetizione del parametro difforme, gli esami microbiologici e le analisi di revisione e analisi chimiche. Tutto questo a favore del consumatore. Il decreto-legge in esame, reintroducendo azioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo nei confronti dei produttori e trasformatori, mette al centro la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute del consumatore e, per essere sufficientemente determinanti e deterrenti, le sanzioni pecuniarie saranno superiori al vantaggio indebito che deriva da pratiche fraudolente e ingannevoli. Inquadrare i reati alimentari nella sfera penale è una scelta italiana molto rilevante, rispettosa per il consumatore. Reputo doveroso perciò ricordare che l'Italia è il Paese più bello del mondo anche e soprattutto per il nostro cibo, frutto della nostra terra, del nostro clima e della nostra passione. Abbiamo perciò il dovere di rispettare i sacrifici delle famiglie italiane che ogni giorno coltivano con amore, cura e fatica i prodotti che portiamo a tavola. Abbiamo il dovere di rispettare le tradizioni che tutto il mondo ci invidia; ci invidia così tanto da volercele declassare, distruggere, rubare o copiare. Abbiamo il dovere di rispettare tutte le tasse che i produttori pagano per far crescere l'Italia. Oggi dall'Europa si impone una disciplina delle abrogazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 27 del 2021, che ha il giusto fine di evitare che rilevanti settori di produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande restino prive di una corretta e doverosa tutela sanzionatoria e amministrativa con pregiudizio, come detto, della salute dei consumatori, che troppo spesso però pretende che vengano rispettati dei regolamenti molto condizionanti, qualitativamente e quantitativamente, mettendo in discussione la storia e la serietà del prodotto italiano. C'è anche lo zampino di qualche burocrate potente, ignorante o servile, che rivendica corrette alcune ridicole scelte, come nel caso del nutri-score che qualche blasonato tecnico italiano, che stranamente passa da ruoli primari in salute a quelli in agricoltura, forse invidiando chi passa dall'economia all'Organizzazione mondiale della sanità, un tecnico che vuole regolamentare il nutri-score per evidenze scientifiche. Non capisce veramente un «cavolo» - è proprio il caso di dirlo in questo caso - o non ricorda nemmeno con quale cibo siano cresciuti lui e i suoi genitori, oppure faccia crescere i suoi figli con tarme essiccate, cibi indefiniti prefritti e bibite gassate. In Italia abbiamo altro, come ad esempio i produttori di lardo di Colonnata, che già da tempo l'Europa voleva mettere in discussione. In Europa però di sicuro non hanno la fortuna di avere la vallata carrarese di Colonnata e non hanno avuto l'intuito di posare il lardo in conche di marmo strofinate con aglio e arricchite di spezie e poi coperte per sei mesi o due anni con un coperchio sempre di marmo. la stessa Europa, che prima ha provato a bandire il prodotto, dichiarando il metodo antigenico, ora dichiara che l'alto contenuto calorico, che era benzina per i lavoratori delle cave, dovrebbe essere un problema proprio per la tabella francese del nutri-score. È uno dei tanti cibi poveri che diventa invece eccellenza: questo è ciò che ci invidiano l'Europa e il mondo, ma non credo che dovremmo sempre dare retta ai burocrati europei, che consigliano poi di fare colazione con una tazza di latte ai piselli e biscotti alla farina di vermi. all'Europa che accetta una bistecca senza carne o un tonno vegetale e che, dopo averci chiesto la lunghezza delle banane, la curvatura dei cetrioli o la lunghezza delle vongole, oggi ci chiede addirittura il vino annacquato. Ma si annacquassero veramente la testa e si rinfrescassero bene, perché non è certo questa la svolta *green*, così come non lo è il nutri-score, se qualifica alcune schifezze alimentari come cibo di serie A, mentre la dieta mediterranea sarebbe un problema. Quando l'Europa chiede agli italiani di tradire l'Italia deve farsi una ragione del fatto che ciò non accadrà mai. Ci sarà sicuramente qualche membro scientifico che cede ai meccanismi europei e alle multinazionali, ma sicuramente non i nostri coltivatori, che non permetteranno mai di cambiare alimentazione ai propri figli. Invece di inventare fesserie, è fondamentale che vengano imposte regole per non far eludere la corretta produzione, come nel caso del pomodoro cinese a tripla concentrazione, che diventa italiano perché - esso sì - innacquato in Italia. più necessario è che l'Europa ci aiuti a combattere l'*italian sounding*. La stessa Europa deve garantire che non arrivi sulla tavola cibo trattato in condizioni igieniche adeguate, in condizioni lavorative disumane oppure ottenuto dallo sfruttamento di uomini, donne e bambini o da animali non controllati e allevati in maniera irregolare. L'Europa deve essere compatta affinché il cibo abbia una filiera sicura e garantita dall'uso di conservanti e diserbanti, dall'uso di concimi e di acqua inquinante e dai terreni dove si produce fino alle fabbriche. Mi chiedo infatti se fuori dall'Italia, dove ogni anno ci sono oltre 900.000 interventi, tra ispezioni e controlli agli alimenti, ci siano gli stessi controlli tecnici e burocratici, se ci siano gli stessi condizionamenti dei grandi distributori,

È auspicabile uniformare in tutta Europa gli obblighi alimentari e sperare che non ci siano bugie, come quando la Francia, approvando una legge sullo spreco alimentare, comunicava che l'Italia era il fanalino di coda. Ebbene, l'Italia è il primo Paese in Europa, basta bugie.

delle carni nei ristoranti, senza ricordare che tra le sue maggiori irregolarità e frodi - i dati sono del 2018 - c'è la presentazione di carni straniere come proprie.

per favorire la scelta dei cibi di serie A, grazie ai profili nutrizionali equilibrati, per l'Italia esso è semplicemente un disonorabile disordine di valutazione. La realtà è che il cibo italiano è imbattibile e solo con la menzogna lo si vuole abbattere. In ogni caso, condivideremo e struttureremo sempre regolamenti che rendano sano un alimento, ma pretendiamo rispetto per la cultura, per le tradizioni e per la filiera di tutto il cibo italiano.

Signor Presidente, gentili colleghi, siamo qui oggi ad apportare le doverose modifiche affinché la sicurezza alimentare sia tutelata sotto tutti gli aspetti giuridici.

si è palesato un testo non conforme a quello presentato alle Camere, che comprendeva l'abrogazione di una serie di divieti nel processo di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti alimentari e le relative sanzioni penali per i trasgressori. Ovvio, quindi, che, in nome di quella sicurezza alimentare di cui spesso ci vantiamo come Paesi ai primi posti su questo tema, il tutto doveva essere prontamente ripristinato. Fortunatamente il sistema democratico funziona in sede sia di disamina delle proposte di legge, che decisionale e il procedimento è trasparente e posto al giudizio di tutti. Difatti, dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* avvenuta l'11 marzo scorso, c'è stata una levata di scudi circa l'imminente pericolo di depenalizzazione di tutti quei divieti presenti negli articoli dell'abrogata legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina della produzione e della vendita di sostanze alimentari. Non è intenzione di questa maggioranza allentare le misure di severità in tema di sicurezza alimentare e lotta alla contraffazione. Tale orientamento è reso esplicito nelle direttive, impartite all'atto della delega al Governo, che salvaguardano le norme penali vigenti. Con il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a convertire il Governo ha rimediato a quel disguido il giorno prima che il provvedimento entrasse in vigore e riaffermato la centralità dell'attività parlamentare. D'altronde, il predetto regolamento europeo recepito rimarca come determinate infrazioni debbano essere punite a livello nazionale in maniera effettiva, dissuasiva e proporzionata, a protezione della salute umana. Tale concetto è ribadito all'articolo 139 dello stesso regolamento. Nelle modifiche apportate dalla Camera dei deputati a questo decreto si ribadisce la linea di severità introdotta applicando le disposizioni del codice di procedura penale nei casi di controllo con prelevamento di campioni e di contestazione degli esiti del controllo. interviene, quindi, sulla disciplina della controperizia e della controversia. Si amplia l'istituto della diffida agli illeciti amministrativi in materia alimentare e si accorciano i tempi per l'adempimento delle prescrizioni. In definitiva, visto il clamore che l'incaglio provocato dal decreto legislativo, qui prontamente modificato, ha suscitato nell'opinione pubblica, soprattutto in una fase della nostra vita così stravolta per via della pandemia in corso, ancora una volta la salute dei cittadini dimostra di essere strettamente collegata alla qualità degli alimenti e alla chiarezza delle informazioni apposte sugli stessi.

Assemblea un ordine del giorno su un prodotto - il miele - fortemente in crisi a causa di pratiche che a oggi eludono i controlli. Si tratta di un tema fondamentale perché attraverso controlli efficaci passano la credibilità delle norme e la loro corretta applicazione; in questo caso passa la certezza della qualità alimentare. Teniamo alta l'attenzione nel campo dell'agroalimentare per continuare a esaltare i nostri prodotti in ambito internazionale, affinché il *made in Italy* mantenga quel valore aggiunto riconosciuto da tutti nel mondo.

però è di estrema importanza, perché di fatto si occupa dell'armonizzazione e dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare. Forse sarebbe necessario che ci soffermassimo a fare una riflessione sul fatto che i provvedimenti dovremmo assimilarli, conoscerli e approfondirli di più, confrontandoci ed eventualmente apportando anche le modifiche necessarie rispetto a quello che è già accaduto

Signor Presidente, cari colleghi, com'è emerso nel corso della discussione, stiamo ragionando di un decreto legislativo, il n. 27 del 2021, che all'articolo 18 ha sostanzialmente abrogato una serie di disposizioni con effetto dalla sua entrata in vigore, cioè dal 26 marzo. Questo decreto legislativo (quindi un atto del Governo) ha inciso sull'elenco di una serie impressionante di norme che sanzionavano,

regole dettate per garantire la salubrità e la genuinità di sostanze alimentari e di bevande. In sostanza, tale decreto legislativo ha cancellato la tutela penale in Italia in materia di sicurezza alimentare e, ciò che è più grave, lo ha fatto con un eccesso di delega, perché, come ha segnalato la Corte di cassazione, ufficio del massimario, nella sua relazione del 17 marzo,

tutti i partiti che oggi fanno parte anche di questa maggioranza, oltre alla Lega e a Forza Italia. Nessuno, però, si è presentato in quest'Aula per spiegare la ragione di tale gravissima forzatura. è difficile credere che si sia trattato soltanto di uno svarione o di una svista. Si è trattato di qualcosa di molto più grave. court* tutte le norme penali che tutelano la salubrità dei nostri alimenti in Italia non può essere soltanto il risultato di una svista. *(Applausi)*. È sicuramente il risultato di un disegno,

su quanto avvenuto e, invece, abbiamo assistito soltanto a un assordante silenzio. Per fortuna, interviene questo decreto-legge, che ripristina tutte le fattispecie sanzionate penalmente agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962,

sul motivo per cui oggi ci troviamo qui a eliminare questo incredibile errore del Governo precedente e poiché nessuno ha ritenuto di dare spiegazioni

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la conversione del decreto-legge n. 42, che siamo chiamati a portare a termine oggi, fa chiarezza e, in qualche misura, dà anche risposte alle questioni poste dal collega sugli obiettivi per i quali, in termini di qualità delle produzioni alimentari del nostro Paese, abbiamo lavorato in questi anni. La qualità dei prodotti, la sicurezza, la salubrità, la volontà di dare al cittadino-consumatore tutti gli elementi per giudicare e scegliere con cognizione di causa la trasparenza sull'origine, sui contenuti e sui processi produttivi sono da sempre al centro dell'azione che il nostro Paese e il nostro mondo agroalimentare hanno posto in campo per ciò che riguarda il cibo, le bevande e tutte le produzioni destinate all'uomo e agli animali.

ci fu una levata di scudi da parte di tutto il mondo che si occupa di qualità agroalimentare. Si gridò, com'è stato fatto qui, a intenzioni equivoche e al gioco sporco, a una norma che di fatto sconfessava la politica sulla quale abbiamo lavorato in questi anni e di cui ho parlato prima. Cos'è successo?

i presupposti per una vera deterrenza, distinguendo tra reati penali e reati sanzionati amministrativamente, nonché a rafforzare il principio di proporzionalità e di chiarezza,

È successo che sullo stesso provvedimento, in sede di Conferenza Stato-Regioni, si è richiesta l'integrazione di tutta una serie di ulteriori abrogazioni come condizione per l'intesa. Probabilmente sottovalutando la portata di quelle stesse abrogazioni, quel testo è stato fatto proprio dal Governo in sede di emanazione del decreto legislativo definitivo.

bevande privati di elementi nutritivi o mescolati con alimenti di qualità inferiore. Venendo meno quel divieto, era possibile farlo. prevedevano il divieto di commercializzare prodotti che fossero in cattivo stato di conservazione, che avessero cariche microbiche superiori ai limiti, che fossero insudiciati o invasi da parassiti o che contenessero residui di prodotti permessi per l'agricoltura, ma tossici e vietati sugli alimenti. Tutto questo (con le relative sanzioni) rischiava di essere cancellato. Ripeto - e credo di poterlo dire senza tema di smentita - che in sede di Conferenza Stato-Regioni questo è stato richiesto come condizione per l'intesa delle Regioni: sicuramente è stata una svista, un errore a cui il Ministero giustamente ha subito posto rimedio con il decreto-legge oggi alla nostra attenzione. Nel percorso di conversione alla Camera sono state inserite alcune norme relative al tema delle controperizie per il campionamento

complessivamente non solo un atto dovuto, ma un buon provvedimento, che introduce norme buone e che ne fa rivivere alcune di cui, allo stato dell'arte, abbiamo assolutamente bisogno. Alla Camera è in corso di attuazione un provvedimento che riscrive tutto il quadro dei cosiddetti agroreati. Credo sia una cosa buona,

dovuto: sicuramente, alla salute degli italiani e a chi crede nella qualità delle nostre produzioni; alla trasparenza che i cittadini italiani ormai si sono abituati a pretendere da tutte le produzioni agroalimentari che arrivano sulle loro tavole; tavole; alla legalità, perché, quando ci sono comportamenti equivoci, dietro c'è sempre il rischio di sacche di illegalità pesante; alla reputazione di questo Paese,

varato dal Governo il 20 ottobre 2020, inviato alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni, non vi era assolutamente alcuna traccia - né poteva esserci - dell'abrogazione di una serie di articoli della legge n.

proprio per il lavoro che sia la Commissione agricoltura, sia le altre Commissioni che hanno inviato il proprio parere hanno fatto in questi anni per la difesa della nostra agricoltura e della sicurezza alimentare. Quando appare questa richiesta?

*(Applausi)*. Le associazioni dei consumatori e del mondo agricolo sono immediatamente intervenute e questo è un fattore importante, perché si sono trovate

della nostra agricoltura, del mondo dell'agroalimentare e dei cittadini.

sull'etichettatura e le iniziative che spesso dobbiamo fare, anche a livello europeo, proprio per difendere la sicurezza alimentare e soprattutto la grande qualità del nostro cibo. Guardate che

messa in commercio e la vendita di sostanze alimentari private dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore, e quindi di contraffazione, oppure in cattivo stato di conservazione

quindi che il Coordinamento interregionale, che si è reso protagonista di quel parere condizionato, si sia reso conto di quale grave danno

la sicurezza alimentare, cioè l'esigenza igienico-sanitaria di consumare sulle nostre tavole prodotti sani, ed è questo un tema ampio, su cui tenere costante l'attenzione. Non è errato quindi affermare che il decreto-legge n. 42 del 2021 mira a tutelare il rispetto di importanti norme dettate per il benessere della collettività. Lo scorso marzo, quando è stato approvato il decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale, mi sono allarmata: come sarebbe stato possibile in poco tempo fare *tabula rasa* di decenni di legislazione, che negli anni si è dimostrata efficace e deterrente contro le frodi alimentari, garantendo a noi sicurezza e salute, senza pensare a un provvedimento alternativo e altrettanto efficace? Difatti, qualche giorno dopo, è seguita l'approvazione del decreto-legge in discussione oggi, che appunto evita l'abrogazione di queste importanti disposizioni di natura sanzionatoria. Ecco perché la materia oggi in discussione è importante: in un Paese con un "*made in*" conosciuto in tutto il mondo e con il maggior numero di prodotti con marchio di qualità (DOP, DOC, IGP, IGT e STG) è fondamentale possedere un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera dell'agroalimentare. solo qualche numero: i dati emersi dall'analisi condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare evidenziano come i cibi provenienti da fuori

significa che l'industria alimentare delle bevande italiane, che - ricordiamolo - è il secondo settore nazionale e che tra mercato interno ed estero produce un volume di consumi che vale 225 miliardi l'anno, ha fatto della sicurezza alimentare un fiore all'occhiello, inserendola completamente all'interno della filiera produttiva come condizione imprescindibile.

in sicurezza e qualità dei prodotti, in investimenti di ricerca e sviluppo, e un miliardo di euro per le analisi di autocontrollo con 85.000 addetti impegnati ogni giorno in attività di analisi e controllo di sicurezza e qualità. La nostra sicurezza in materia è ulteriormente tutelata anche grazie al lavoro svolto quotidianamente dal dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf). Tra le molte attività dell'organo di controllo del Ministero per le politiche agricole e forestali segnalo l'importante ruolo nel contrasto delle pratiche sleali, il quale costituisce un importante contributo alla tutela del comparto agroalimentare. Possiamo quindi affermare con molta chiarezza che l'Italia ha fatto della sicurezza alimentare parte della realtà produttiva, storica e culturale che si contraddistingue in tutto il mondo. Sul tema dei controlli, anche se molti sono stati i progressi fatti negli anni per armonizzare al meglio il sistema, credo sia però opportuno un ulteriore sforzo verso la loro piena centralizzazione, creando un registro unico dei controlli, rendendo così più efficiente il lavoro svolto dagli operatori ed evitando ridondanze organizzative. Per questo motivo, scongiurando definitivamente oggi l'effetto abrogativo delle disposizioni sanzionatorie in materia agroalimentare, chiedo però di rinnovare l'impegno a tutela dei consumatori e soprattutto del settore dell'agroalimentare nel combattere qualsiasi tipo di attacco volto a ledere gli interessi del *made in Italy*. Penso alla contraffazione dei marchi, alla falsa indicazione del *made in*, alle forme di etichettatura ambigue. Cito qualche numero: nel periodo 2008-2018, 542 milioni sono stati i pezzi sequestrati, per un valore complessivo di oltre 5,5 miliardi di euro. Tutelare il *made in* vuol dire anche spingere sempre di più su sistemi di tracciabilità dell'intera filiera, per due ordini di motivi: il primo è legato alla sicurezza dei consumi, cioè dare la consapevolezza al consumatore di cosa sta acquistando; il secondo è il seguente: legare ancora di più il prodotto al proprio territorio, territorio, alla sua storia e alla cultura. Infine, chiedo ancora una volta di contrastare in sede europea la possibilità di applicazione del nutri-score, che come Gruppo Forza Italia abbiamo più volte contrastato: l'etichettatura a semaforo metterebbe a rischio la produzione italiana, creando falso allarmismo per il consumatore nei riguardi dei prodotti tipici della dieta mediterranea, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità, nonché imitata - con scarso successo, in realtà - in tutto il mondo. La nostra missione dev'essere quella di tutelare gli operatori virtuosi che quotidianamente rendono grande il *made in Italy* alimentare in Italia e nel mondo, evitando che il consumatore possa essere influenzato da esternalità che mirano semplicemente a far fuori un *competitor*, appunto l'Italia, che da anni conserva il primato nel settore. Concludo dicendo che attraverso questo decreto-legge si consente al sistema agroalimentare italiano di conservare il ruolo apicale nel mondo per gli *standard* di sicurezza alimentare adottati. Annuncio quindi il voto favorevole di Forza Italia. rappresentanti del Governo, colleghi, l'Atto Senato 2201 concerne la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che disciplina la sicurezza alimentare. Già il titolo dovrebbe far capire che si tratta di una fattispecie di estrema rilevanza per il settore di interesse, l'agroalimentare italiano, perché la sicurezza alimentare è un tema che da noi è molto sentito, ma in altri Paesi evidentemente no. Non credo serva essere patriottici per considerare l'Italia uno dei Paesi in cui si mangia meglio al mondo e dove si producono alcuni tra i migliori prodotti, di qualità superiore in assoluto in ambito alimentare. Questo avviene sia perché il prodotto di base è di qualità molto elevata, sia perché i nostri artigiani, a mio avviso, meriterebbero il titolo di maestri per la capacità di lavorare le materie

mi trovai con un allevatore che aveva due capi contagiati dall'anemia infettiva equina, per cui emanai un provvedimento restrittivo, che mi insegnò una cosa molto importante: che a parole sono tutti a favore della sicurezza alimentare e tutti vorrebbero che fosse un elemento imprescindibile nella produzione dei nostri prodotti tipici; poi però, nei fatti, non tutti sono disposti a comportarsi coerentemente con questa enunciazione. Ricordo, sempre parlando per esperienza diretta, che l'allevatore, anziché adeguarsi al mio provvedimento, tentò di ribellarsi in ogni modo e addirittura arrivò a chiamare «Le Iene». Potete immaginare quante centinaia di *email* Rispondevo a tutti con tre semplicissime righe: ma per la vostra tavola o per quella dei vostri figli preferireste che arrivasse una bistecca controllata o non controllata?

che ha un costo di produzione di 1,24 euro, quando in realtà credo che in Italia non si potrebbe realizzare un prodotto analogo nemmeno spendendo il triplo; che vorrebbe vietare ai nostri anziani di produrre direttamente per l'autoconsumo negli orti e che però consente l'importazione di prodotti che nella loro filiera non hanno alcun tipo di controllo relativamente non solo alla loro qualità,

nel circolo dell'alimentazione e della vendita. Mi riferisco a tutte quelle verifiche che diamo per scontate, perché implicite nel nostro sistema, ma che scontate non sono e che purtroppo rischiano non solo un settore che è già pesantemente danneggiato, per tutte le contraffazioni alimentari e per il falso *made in Italy*, ma anche di penalizzare direttamente i nostri produttori, che naturalmente tendono ad adeguarsi, invece, a queste prerogative. Come dicevo prima, voglio porre l'accento su quanto disciplinato direttamente nel provvedimento e, per evitare di dimenticare qualcosa, leggo testualmente quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge, l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio riguardo all'igiene e alle sostanze alimentari. A tal riguardo, degna di mantenimento è la legge n. 283 del 1962 che, all'articolo 5, vieta espressamente l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano state private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate, oppure in cattivo stato di conservazione, o con cariche microbiche superiori al limite stabilito, oppure con l'aggiunta di additivi non autorizzati. In sostanza, si tratta dell'essenza dei nostri prodotti che rischiava di essere minacciata - appunto - dall'abrogazione di un testo che, a mio avviso, dovrebbe essere alla base di ogni produzione di qualità mondiale, ma che di fatto in altri Paesi del mondo non si riscontra, facendo sì che le nostre tavole fossero raggiunte da prodotti di qualità estremamente inferiore a quella a cui siamo abituati. Inoltre, i nostri produttori si potevano trovare di fronte a una concorrenza sleale come quella che evidentemente rappresenta chi riesce a realizzare il prodotto finale senza nessuna delle condizioni a cui invece dobbiamo sottostare noi, evidentemente andando a creare un danno per la nostra economia. Ritengo giusto, quindi, che all'articolo 6 rimanga la previsione di una rilevanza anche penale relativamente a queste fattispecie, perché sappiamo bene che la sanzione amministrativa già di per sé non sarebbe un deterrente sufficiente, poi in molti casi sarebbe anche difficile da applicare. Pertanto, la rilevanza penale per chi minaccia la sicurezza alimentare delle nostre tavole, a mio avviso, è un obiettivo

chi eventualmente introduce questi alimenti da noi, non rispondendo a quelle caratteristiche fondamentali, ma anche evitare l'introduzione di tali prodotti, perché solo questo garantisce il nostro sistema produttivo e agroalimentare

la tutela del *made in Italy,* del nostro sistema produttivo, del nostro artigianato e del nostro allevamento potrebbe essere altrettanto fondamentale del *recovery plan,* che indichiamo in questo momento come unica strada possibile per uscire dalla crisi, ma che, a mio avviso, potrebbe avere un'alternativa altrettanto valida, valorizzando quello che abbiamo sempre dato per scontato, ma che invece evidentemente scontato non è. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci accingiamo a votare un provvedimento esaminato in prima lettura alla Camera e in seconda qui al Senato, che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare ed è volto a circoscrivere l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, ovvero l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principi illeciti amministrativi. Il provvedimento salvaguarda il *made in Italy* ed è importante perché ci troviamo di fronte a una vera e propria transizione nutrizionale tale per cui, grazie a mezzi chimici sempre più sofisticati, riusciamo a diagnosticare abbastanza presto e accuratamente malattie legate al tipo di alimentazione che impatta sulla nostra salute. Per fortuna, l'Unione europea si è fornita nel tempo di regolamenti idonei per la produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e di origine animale. Infatti, già alla fine degli anni Novanta in Europa si andò formando una coscienza diffusa sui rischi alimentari e sulle possibili contaminazioni chimiche, biologiche e fisiche. In quegli anni, fecero scandalo le frodi alimentari, come le adulterazioni e le sofisticazioni, perciò i primi anni del Duemila furono caratterizzati da un'intensa attività legislativa sull'igiene dei prodotti e degli alimenti di origine animale, sui controlli ufficiali degli animali destinati al consumo umano e sulle condizioni di salute dell'ambiente degli animali stessi. Infine, nel 2002, venne istituita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge bene il suo lavoro. Tutto ciò, tuttavia, oggi rischia di essere vanificato dalle logiche di mercato che immettono alimenti di origine vegetale ed animale dei Paesi extraeuropei che non hanno le stesse normative di tutela. Non voglio parlare dei prodotti provenienti dai Paesi africani o dai Paesi asiatici, ma mi soffermo solo su quelli statunitensi. Basti pensare che, nell'ambito dei prodotti alimentari, nell'Unione europea vige il principio di precauzione, mentre negli Stati Uniti no: un alimento è sicuro fino a prova contraria. Purtroppo, però, alcune sostanze chimiche presenti nei prodotti danno i loro effetti nel tempo, basti pensare alla presenza di glifosati nel frumento, che invadono i nostri mercati e che si mescolano nel nostro frumento di qualità migliore e di salubrità indiscussa. indiscussa. In questo scenario, andrebbero aggiunte anche le patologie che si manifestano nel tempo e che certi studi ancora stanno verificando. Mi riferisco, ad esempio, ai casi di celiachia correlati all'uso di glifosati. Dopo questa dovuta cronistoria sulla sicurezza alimentare, definiamo lo scopo del provvedimento in esame, ovvero quello di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale ed amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori. alla Camera sono stati inseriti due aspetti inerenti alla controperizia e alla controversia in un provvedimento che comunque mira a circoscrivere l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo del 2 Per quanto attiene le competenze della Commissione agricoltura, di cui mi onoro di far parte, ancor di più da siciliana e da donna del Sud, va sottolineato anzitutto l'articolo 1, che interviene sul già citato articolo 18 e che incide sull'elenco di abrogazioni per circoscriverne la portata ed in particolare impedire le abrogazioni dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande. L'articolo 18, infatti, dispone l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 30 aprile 1962, quindi una legge di sessant'anni fa, obsoleta, per cui è necessaria una chiave di interpretazione calata nella contemporaneità, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principi illeciti amministrativi relativi all'impiego o alla somministrazione di sostanze alimentari e di bevande, sanzioni che sono state comunque reintrodotte grazie al nostro lavoro Questo provvedimento è importante proprio perché va ad individuare le Autorità atte a organizzare o a effettuare controlli ufficiali, comprese le attività nei diversi settori che riguardano gli alimenti, la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità in tutte le diverse fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, ma anche la messa in commercio di sostanze alimentari con imballaggi colorati comunque non autorizzati. Mi avvio alla conclusione, Presidente, ripercorrendo sia il concetto della transizione nutrizionale alimentare, sia il concetto della transizione ecologica, l'uno imprescindibile dall'altro, di dimensioni - soprattutto quest'ultimo - epocali, a cui tutti siamo tenuti a partecipare e che rappresenta un'occasione unica per poter intervenire con un approccio olistico che possa coniugare salute e rispetto dell'ambiente, un'opportunità per migliorare la vita dei cittadini, perché a noi sta a cuore il loro benessere. L'obiettivo finale è la sicurezza alimentare per il benessere della collettività. Molti prodotti, infatti, contengono ingredienti dannosi per la salute dei nostri cittadini,

che possono causare alcuni prodotti alimentari, su cui bisognerebbe, per una maggiore trasparenza, introdurre un'etichetta quanto più possibile colma di informazioni sui prodotti, ma corredata anche, a mio avviso, da un *logo* a connotazione regionale, che possa limitarne la contraffazione. Concludo proprio con questo auspicio, nel ribadire il voto favorevole del Gruppo del

non c'è pace per il patrimonio culturale della città di Napoli, troppo spesso esposto al rischio di dispersione, se non di vera e propria distruzione. Mi riferisco al patrimonio immobiliare, non meno che alle opere di interesse storico-artistico, e così pure all'artigianato artistico. Che dire della svendita del palazzo del Monte di Pietà a Spaccanapoli; la cordata guidata da Michele Amoroso avrebbe raggiunto un accordo con la proprietà, passata da circa venti anni da un istituto di credito di diritto pubblico, il Banco di Napoli, ad uno di diritto privato, Intesa Sanpaolo, che mentre si autocelebra per le gallerie d'Italia, dimostra di non avere compreso il valore di quello scrigno di storia e di arte, identitario per tutti i partenopei, che è il Monte di Pietà. Con i colleghi di L'Alternativa C'è nell'interrogazione presentata in aprile abbiamo ipotizzato che lo Stato e gli enti locali esercitino la prelazione e il palazzo, compatibilmente con la sua dignità, possa accogliere istituti di istruzione universitaria, come la Scuola superiore meridionale o un archivio dei più importanti. Due settimane fa la commissione cultura del Comune ha finalmente battuto un colpo e vedremo cosa porterà il futuro. Restando in tema di palazzi storici, è del 3 maggio la notizia del principio di incendio sviluppatosi in un magazzino al quarto piano di Palazzo Reale. Ha avuto un esito più felice invece la battaglia per salvare la sartoria teatrale di Vincenzo Canzanella che, sfrattata dai locali di Sant'Eligio, anche grazie all'impegno dell'onorevole Maria Muscarà, trasferirà a Bagnoli la sua sede operativa. Un'esposizione dello straordinario campionario di opere realizzate in circa cinquanta anni di attività deve però restare a Napoli e c'è da augurarsi che la proposta di allocarla nei locali sottostanti la chiesa di San Francesco di Paola trovi orecchie disposte ad ascoltare. Più scabrosa delle precedenti è infine la vicenda delle 400 opere di proprietà comunale custodite nel deposito sotterraneo del Museo Civico di Castel Nuovo, in ambienti malsani, danneggiate da ultimo dalla pioggia dello scorso novembre. All'intervento di semplice messa in sicurezza promosso dal Comune con una somma modesta dovrebbe fare sponda il trasferimento coatto in un museo disposto dal soprintendente grazie all'applicazione dell'articolo 43 del codice dei beni culturali. A causa delle riforme Franceschini però la soprintendenza non ha più alcun rapporto con i musei del territorio e i loro depositi il soprintendente di Napoli è un dirigente di seconda fascia, mentre i musei dipendono dalla direzione regionale musei, che fa capo alla direzione generale musei o addirittura sono istituti autonomi, come Capodimonte, retti da direttori generali. La tutela del patrimonio culturale italiano è dunque resa impossibile tecnicamente dallo stesso Ministero preposto a realizzare l'articolo 9 della Costituzione, un Ministero suicidato dal suo eterno titolare e dai cortigiani di cui si è circondato, eterodiretti l'uno e gli altri da potentati economici e massoneria deviata. Mi appellerei al Presidente della Repubblica, se non nutrissi dubbi anche sull'efficacia di un simile appello.

intervengo in quest'Aula per sollecitare il Ministro dell'economia e delle finanze a venire a riferire in Parlamento sullo stato di avanzamento dell'importante, quanto delicato, *dossier* di Autostrade per l'Italia. Dopo il grande lavoro fatto, ora è giunto il momento di portare a casa il risultato, togliendo le nostre autostrade dalle mani di chi ha fallito e facendole tornare sotto la gestione pubblica. A luglio 2020 si è definita la strada per chiudere questa vertenza, non con la revoca per cui ha sempre lottato il MoVimento 5 Stelle e che non abbiamo potuto ottenere, non per colpa nostra, ma perché era necessaria una maggioranza in Parlamento che non c'è stata data, né con il Governo Conte I, né con il Governo Conte II. Per questo abbiamo accettato, seppur con fatica, la soluzione di compromesso del subentro di Cassa depositi e prestiti nella quota di Atlantia SpA, ma le notizie delle ultime settimane non sono per nulla confortanti: c'è una grande incertezza. Soprattutto, riteniamo inaccettabile la decisione interna ad Autostrade per l'Italia (Aspi) di aumentare i già esorbitanti stipendi dei massimi vertici, il tutto - pare - con l'avallo del consorzio subentrante, tra cui appunto Cassa Questo non va bene. Le famiglie delle vittime meritano giustizia, i genovesi meritano giustizia, tutti gli italiani meritano giustizia e autostrade sicure. Manca solo l'ultimo miglio, con la cacciata di coloro che, per bramosia di denaro, hanno lasciato nell'incuria il ponte di Genova fino a farlo crollare, signori che oltretutto, in questi mesi di limbo, hanno continuato a incassare una marea di soldi. Venga il ministro Franco a riferire in Parlamento nelle modalità che riterrà più opportune. Il MoVimento 5 Stelle, dal canto suo, chiede invano da almeno due mesi la presenza del Ministro in diretta televisiva in un *question time.* La pazienza è abbondantemente finita e per questo chiediamo che la Presidenza del Senato si faccia parte attiva per consentire a questo ramo del Parlamento, e quindi a tutto il Paese, di essere aggiornati su questo importantissimo *dossier*. *(Applausi)*.

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune settimane or sono ho incontrato una delegazione dei ristoratori della mia zona, ristoratori che, come potete ben capire, sono allo stremo, in una condizione di grave prostrazione, non solo economica, ma anche psicologica. Da quell'incontro, oltre ad emergere l'ovvia necessità di lavorare immediatamente, necessità cui finalmente il Governo ha risposto proprio ieri con un decreto che è stato da noi fortemente voluto, è emersa anche un'altra cosa e cioè che i ristoratori non possono restare in balia

Come si fa a dare questa possibilità? Quest'anno abbiamo avuto il Covid-19; potrebbe esserci una recrudescenza l'anno prossimo, potrebbe arrivare qualche altra malattia.

per aiutarlo. Ad esempio, ci sono dei sistemi di filtraggio dell'aria come sugli aerei? Usiamoli, diamo la possibilità ai ristoratori di usarli attraverso opportuni incentivi fiscali.

anno e renderle maggiormente fruibili e utilizzabili dagli stessi imprenditori. Quindi, signor Presidente, al compiacimento per le nuove disposizioni del Governo Draghi, uniamo il grido di dolore e l'immediata e fattiva richiesta di un nuovo ripensamento per la categoria.

Sacella, parroco di una comunità di 600 parrocchiani a Torre Maina, nel Comune di Maranello, in Provincia di Modena. Don Pierino Sacella, che indossa il cappello da alpino ed è stato cappellano dell'Accademia militare di Modena e che io ho avuto modo di conoscere personalmente,

(da sua mamma, *in primis*, e da suo papà): egli è un uomo della natura, un cacciatore rispettoso dell'ambiente e delle leggi. Don Pierino, purtroppo, è stato vittima di vergognose azioni di terrorismo animalista. Il paese,

Lo svolgimento della messa dell'Immacolata è stata ostacolata da questi facinorosi con degli *slogan* ingiuriosi e un presidio verbalmente violento è stato attivato durante la messa di Natale, quasi a impedire ai fedeli di entrare in chiesa: se ti troviamo in campagna, non sarai protetto dalle mura della chiesa. Come avete capito, i fatti non sono recenti perché il Covid non li avrebbe permessi, però è recentissimo

non nuove nell'espletare atti violenti e vandalici che lo Stato deve combattere con le dovute energie. Al povero don Pierino Sacella, prete e cacciatore, alla solidarietà che gli è stata trasmessa da tutti i suoi parrocchiani aggiungo anche la mia e quella di tutte le persone perbene. E lo faccio a maggior ragione oggi, perché voglio ricordare che questa mattina

Se qualcuno pensa di usare l'arroganza e la violenza per imporre sbandate filosofie animaliste lesive delle nostre culture rurali sta sbagliando e i parrocchiani di Torre Maina saranno allora destinati ad aumentare a dismisura.